conti. È importante contestualizzare l'ingresso nella normativa italiana della segnalazione d'irregolarità, perché nasce praticamente nella fase in cui il Parlamento italiano ha tentato di dare risposta alla battaglia contro la corruzione, che - ahimè - vede ancora l'Italia sconfitta dal punto

Ciò che cambia è il contesto generale. Il pregio del disegno di legge, di cui ha avuto molta cura il relatore, qui presente, che ringrazio per l'attenzione che ha prestato a tutte le osservazioni anche informali che abbiamo svolto in Commissione prima e dopo le audizioni,

di istituto autonomo con una legge che lo regolamenta e questo è un fatto che aiuterà anche la diffusione nel Paese di una nuova cultura.

e la delazione. No, esiste un'altra fase, un'altra possibilità di essere pubblico dipendente o collaboratore dell'amministrazione o anche dipendente privato in settori in cui si annida spesso la corruzione, come i settori privati che esplicano servizi per la pubblica amministrazione e quindi vivono vivono di soldi pubblici. Esiste un'altra possibilità e, cioè, la segnalazione di una persona corretta che vede qualcosa che non va nell'ambito della propria organizzazione aziendale o nell'ambito della pubblica amministrazione.

si risolve affrontando il tema e stabilendo che non tutto è denuncia all'autorità giudiziaria, non tutto ha bisogno di una denuncia al giudice giudice o alla Corte dei conti, cioè al giudice che guarda ai conti pubblici, ma che c'è uno spazio autonomo, occupato dal punto di vista del controllo e dell'erogazione delle sanzioni dall'ANAC, che prevede segnalazioni fatte

il pubblico dipendente è già obbligato a denunciare reati. Qui non si tratta di un reato *tout court*; non è il caso del dipendente che vede commettere un reato di altra natura o che occasionalmente viene a sapere di qualcosa e riferisce. Si tratta di segnalazioni che hanno

Qual è, dunque, l'obiettivo dichiarato della norma, che oggi è scritta molto meglio? La prevenzione della corruzione; quindi nessun allarme deve ostacolare questo percorso, che è innanzitutto culturale. Non dobbiamo essere allarmati dal fatto che in una pubblica amministrazione un

il disegno di legge in esame, che riguarda la segnalazione anonima di fatti illeciti nella pubblica amministrazione o in aziende che abbiano rapporti con il perimetro pubblico, ha registrato la netta contrarietà del Gruppo Forza Italia. La 1a Commissione del Senato ha diffusamente modificato quel testo, ma non ne ha eliminato le criticità che, a nostro avviso, dopo quasi due anni, non solo permangono tuttora, ma si sono addirittura Vale la pena segnalare subito che una normativa analoga a quella al nostro esame è stata introdotta nel testo unico bancario dal legislatore (articolo 1 del decreto legislativo del 12 maggio 2015, n. 72) in recepimento della direttiva 2013/36/UE. Così come va rilevato che il testo unico sulla finanza è stato integrato mediante la legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea, secondo semestre) in attuazione della direttiva citata. La differenza rispetto al testo in esame è però molto semplice. In quei testi viene garantita la riservatezza dei dati personali del segnalante, ma anche quella del segnalato, che viene sempre ritenuto «presunto responsabile» della violazione, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento giudiziario. Al contrario, con l'impostazione data dal disegno di legge in esame si rischia di lasciare su una graticola mediatica colui che viene segnalato, senza potere adottare misure contro il segnalante, che si rivelasse in mala fede, nemmeno a procedimento concluso. Lo scopo di una legge non può quindi essere solo quello di incrementare il numero delle segnalazioni di abusi o illeciti nel perimetro pubblico. La segnalazione deve essere un atto certamente tutelabile, se al contempo si tutela anche il segnalato, che, fino a prova contraria, deve essere considerato «presunto innocente». Il rischio è, appunto, quello di una lunga esposizione mediatica per colui che viene segnalato, mentre al segnalante sono garantiti l'anonimato e l'intoccabilità sino alla fine dei procedimenti. Non vi sono provvedimenti a carico di chi avesse eseguito una segnalazione in malafede, per vendetta o ritorsione, o qualsivoglia altro motivo. Si dovrebbe allora attendere un eventuale procedimento per i reati di calunnia o diffamazione nei confronti del segnalante. Va detto che, peraltro, si tratta di reati - la diffamazione, la calunnia - sempre difficili da dimostrare. E comunque bisognerebbe attendere un *iter* processuale successivo a quello del proscioglimento della persona segnalata. Noi siamo convinti che i rappresentanti politici non debbano oggi fare una inutile gara a chi è il più onesto. L'onestà è, ovviamente, un prerequisito per chi voglia fare politica o per chi voglia occuparsi di gestire, in qualsiasi modo, la cosa pubblica. Su una normativa di questo tipo era però necessario trovare un testo più largamente condiviso dalle diverse forze politiche. Ma soprattutto era necessario un articolato di legge equilibrato e più garantista, coniugandolo con la necessità di combattere ogni forma di reato in danno dell'interesse pubblico. Non si possono non evidenziare i problemi di carattere pratico che la novella proposta porta con sé, come quello di dimostrare la buona fede o la malafede. Così come difficili da dimostrare rimangono il dolo o la colpa grave di chi effettui segnalazioni infondate. Un tema come questo, che interessa noi tutti, deve poggiare su termini di diritto e non su disposizioni alquanto vaghe e dai contorni indefiniti. Il problema non si risolve quindi con una modifica di questo tipo dell'articolo 54-*bis* del testo unico sul pubblico impiego e delle norme ad esso collegate. Anche prendendo spunto dalle regole adottate da altri Paesi, dove il *whistleblowing* funziona e aiuta a scoprire i reati contro la pubblica amministrazione, bisognava quindi modificare la normativa esistente, rendendo più facile perseguire gli illeciti in qualsiasi modo collegati a denaro pubblico. Ma bisognava farlo rispettando le elementari regole del diritto, che prevedono la presunzione di innocenza fino a prova contraria, anche di chi viene denunciato da un segnalante anonimo. In tal senso, riteniamo che si debba tener conto di tutte le implicazioni che comporta il nuovo articolato, sia nel settore pubblico che in quello privato che abbia rapporti con le pubbliche amministrazioni per appalti, subappalti o concessioni. Altrimenti si rischia, come appunto stiamo facendo, di mettere in piedi una normativa molto pericolosa, che oltretutto potrebbe essere censurata dalla Consulta, considerati i forti dubbi di costituzionalità che emergono alla luce del principio della presunzione di non colpevolezza

Signor Presidente, la corruzione è una cosa bruttissima, è una metastasi che nel Paese aumenta i costi dei servizi pubblici del 40 per cento, che uccide le aziende sane, che affossa il merito e che porta ogni anno almeno 60-70 miliardi di costi in più (le valutazioni sono diverse nei diversi settori). Certo è che, proprio grazie alla corruzione, abbiamo appalti che lievitano, soprattutto quando, sotto una certa cifra, non è necessario il bando di gara, ma basta il confronto tra le offerte. La corruzione, quindi, è quasi endemica. Tra l'altro, noi facciamo una figura pessima, perché, secondo la classifica di Trasparency International, International, siamo al 60º posto nel mondo e siamo terz'ultimi in Europa per trasparenza. Lo stesso Papa Francesco parla di corruzione ovunque, ma la corruzione è anche in Vaticano. La corruzione è qualcosa che peggiora lo Stato, le prospettive e anche le speranze; diventa endemica nelle istituzioni, come abbiamo visto più volte. L'abbiamo visto tra Buzzi, Carminati, Raggi e Marra: anche chi voleva essere esempio di trasparenza e correttezza ha dato poi il suo peggio. Ricordo un articolo del 1955 su «L'Espresso», che parlava di capitale corrotta e nazione infetta. si è cercato di fare molto, ma spesso ottenendo dei risultati deludenti. A volte, i controlli sui controlli hanno

è tutta teorica. E allora che fare per combattere la corruzione? Cicerone diceva che l'onesto è l'uomo degno di onore. Per avere onore non c'è legge, non c'è deterrenza, non c'è sanzione perché l'onore rientra in una sfera molto più intima

questi gendarmi di controllo c'erano. C'erano le famose spie, quelle che fanno magari il filmino quando un senatore vota per il collega che sta due banchi sotto che però,

più chiara da capire. Chiedo, pertanto a chi fa tanta esaltazione dell'onestà: dov'erano i colleghi del Movimento 5 Stelle, quando io stessa venivo diffamata con notizie non vere, e loro lo sapevano però nessuno nessuno azzardava una difesa; quando venivano espulsi altri colleghi con altrettante falsità e nessuno aveva il coraggio di denunciare e di dire che non era vero per paura di perdere la prossima candidatura, una poltrona? Questa Questa è l'onestà dei vigliacchi, è l'onestà che parla di trasparenza ma nasconde i bilanci, che parla di meritocrazia, di *curriculum* inviati e assume parenti,

semplificazione, perché se mettiamo tutto in luce, rendiamo ogni cosa più semplice, più equa, più vivibile. Forse, allora, i cittadini saranno spontaneamente portati a essere anche più onesti. Ho sentito certe sviolinate che mi hanno veramente disgustata, pensando all'incoerenza nelle piccole e nelle grandi cose:

interpretare la legge nel modo più utile e non più giusto. Non bastano sicuramente le leggi:

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è elusivo dell'apparato di garanzie cui tende, in uno Stato di diritto, il processo penale. Dietro il paravento della segnalazione effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, infatti, si cela il tentativo di abbassare la soglia delle tutele che, dinanzi a un'accusa, spettano a ogni cittadino. In questa fattispecie, infatti, la trasmissione della denuncia al giudice penale è solo eventuale: badate che non è un caso limite. È già avvenuto che la sindaca di una grande città avesse trasmesso atti all'ANAC e che questa Autorità si fosse limitata a esprimere un parere invece di ravvisare elementi di sospetto in una determinata nomina, salvo poi accorgersi della cosa in ritardo - quando scoppiò lo scandalo mediatico - trasmettendo gli atti alla competente procura di Roma. Alla faccia dell'obbligatorietà del rapporto in caso di illeciti penali! Dietro lo schermo della segnalazione effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione si cela, quindi, una grande ipocrisia. Per non impegnarsi nel deferimento dei possibili illeciti all'autorità giudiziaria, si crea un apparato sanzionatorio parallelo, che passa per l'amministrazione e arriva all'ANAC, che si riterrà soddisfatto anche solo con un principio di prova, senza sollecitare l'assai più rigoroso scrutinio (indizi chiari, univoci, concordanti) che richiede, appunto, il giudizio penale. In altre parole, tutte le volte che si riterrà non poter provare un episodio corruttivo, sarà assai più comodo attestarsi sull'ipotesi minimale della *mala gestio*, per punire in sede disciplinare - o, peggio ancora, extra amministrativa, grazie alle determine dell'ANAC chi non ha modo di difendersi, rimanendo, appunto, appeso a un filo. Già, perché in una qualche fase del giudizio penale l'imputato giunge comunque a conoscere il nome di chi lo accusa, ne viene a conoscenza. Infatti, uno degli elementi fondamentali della difesa è quello di dimostrare la non credibilità dell'accusatore. Come si fa a ottenere lo stesso risultato in un giudizio amministrativo nel quale questo nome, presto presto o tardi, non salta fuori? L'esigenza sottesa al testo è giusta, ma andava soddisfatta diversamente, senza abbassare il livello delle garanzie. La mia proposta, in sede di esame del disegno di legge n. 19, fu anche più rigorosa. L'emendamento 5.0.302, a mia firma, intendeva punire con l'arresto fino a sei mesi «chiunque pubblica in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, l'identità del segnalante», fino a quando l'indagine preliminare fosse stata in corso. mi mantenevo, non a caso, all'interno del sistema processuale penale, rispettando il punto di equilibrio - ivi previsto - tra le responsabilità di ciascuno: imputato, accusatore, giudice, tutti alla luce del pubblico dibattimento. La Presidenza preferì tuttavia dichiararlo improponibile per dare invece spazio a questo testo che deroga alle garanzie processuali più elementari. Visto che ci siamo, segnalo un'altra anomalia della gestione parlamentare di questo testo, che inizialmente era stato deferito alle Commissioni riunite giustizia e affari costituzionali. Poco dopo il suo arrivo dalla Camera dei deputati, con riferimento espresso a tale disegno di legge i deputati radicali della scorsa legislatura presentarono la petizione n. n. 1.538, che proponeva l'estensione della possibilità di *whistleblowing* anche ai dipendenti dalle Camere. Fu anch'essa deferita alle Commissioni riunite e lì è rimasta, anche dopo che, con decisione discutibile, il disegno di legge passò alla sola Commissione affari costituzionali.

Non si capisce, infatti, perché continuare a escludere, quanto meno dalla normativa Severino già esistente, una nicchia amministrativa che in passato si è segnalata per opacità. ha evaso l'IVA sugli affitti della Camera del 2011 (come accertato dalla sentenza del tribunale di Roma in questa settimana), forse sono tenuti a saperlo anche coloro che gestivano il contratto dal lato dell'affittante. Se il contenuto della petizione fosse stato legge, ce ne saremmo accorti tutti prima e, forse, il discredito per le istituzioni che sopportano il peso di queste situazioni sarebbe stato minore. Ci sono però responsabilità del legislatore: leggi equivoche, contraddittorie e incerte nella loro definizione e tassatività, zone grigie volute o irresponsabilmente determinate. Sono anche alla base di uno stato generale, oltre a essere qualsiasi controllo amministrativo preventivo che, appunto, non agisce in maniera precauzionale, mettendo in discussione - anzi, sanzionando - gli atti amministrativi non conformi alla legge. Ci sono responsabilità degli amministratori, sindaci e Presidenti. Nell'indagine che la Commissione antimafia ha fatto sul Comune di Roma è emersa in maniera chiara l'assenza di qualsiasi controllo interno, qualsiasi *audit* o ispettorato che esercitasse un controllo preventivo all'interno di un'istituzione che, con le sue partecipate, conta circa 60.000 dipendenti. Ci sono però responsabilità anche più generali del nostro Paese, cioè di noi cittadini. È un Paese povero moralmente questo, se deve premiare chi fa solo il proprio dovere. È un Paese povero questo, se deve proteggere coloro che fanno solo il proprio dovere. È un Paese povero questo, che ha bisogno, anche in tempi di pace, di eroi. Signor Presidente, io non mi rassegno. Credo in un Paese in cui ci sono ancora coloro che non si piegano all'omertà, all'arbitrio e alla convenienza personale. Ci sono cittadini e parlamentari che dicono quello che pensano e fanno quello che devono.

vuole essere insensibile rispetto alle esigenze di trasparenza delle nostre attività pubbliche e private come nessuno è certamente insensibile rispetto all'esigenze di tutela di coloro che - doverosamente - segnalano anomalie e patologie nelle pubbliche amministrazioni, così come nelle attività produttive di beni e servizi. Il problema a questo punto è la qualità della legislazione di cui stiamo discutendo, dell'adeguatezza dello strumento che è in discussione ai fini

alle altrettanto evidenti esigenze di stabilità delle attività pubbliche, delle attività delle pubbliche amministrazioni come delle attività economiche. Un potenziale conflitto tra le esigenze di stabilità e quelle di tutela della segnalazione da parte di dipendenti di comportamenti patologici è dato dall'inevitabile possibilità di segnalazioni temerarie che si rivelino, non a prima vista, ma in un tempo differito, assolutamente infondate.

interessati al prodursi degli atti contestati e che verrebbero evidentemente nel frattempo sospesi) e

Ho detto ieri che il testo al nostro esame sembra una traduzione abbastanza diretta delle discipline proprie del sistema di *common law*, che ha tuttavia un ordinamento giudiziario con capacità d'indagine e di decisione sulla base dei precedenti che non si rinvengono nel nostro ordinamento. D'altronde, anche e soprattutto nei sistemi di *common law*, alla fine la trasparenza e la correttezza sono affidate a regole di operatività tanto delle pubbliche amministrazioni quanto delle attività economiche, a regole che determinino una serie di presidi alle anomalie e alle patologie,

comunità di cui facciamo parte, che ci conducono a non accettare la patologia quando la incontriamo e ne veniamo a conoscenza. Credo che i pericoli maggiori impliciti in questo provvedimento riguardino soprattutto le pubbliche amministrazioni. Non dimentichiamo le ragioni della loro persistente persistente fragilità nonostante i tentativi di riforma che sono stati attuati, anche con produzione torrenziale di norme, nel corso degli ultimi Si è più volte riscontrata l'esigenza di introdurre in esse la figura del buon datore di lavoro; non mi riferisco ad un figura specifica, ma ad un ordine delle cose che faccia riconoscere la presenza del buon datore di lavoro oggi assolutamente assente. In questo contesto fragile, nell'assenza del buon datore di lavoro, molto spesso gli ambienti delle pubbliche amministrazioni, a differenza di ciò che accade più diffusamente nella dimensione privata, diventano focolai di frustrazioni, di invidie, di vendette e di gelosie. In ogni caso, sono luoghi nei quali difficilmente viene accettata la promozione altrui, ritenendosi sempre e comunque discriminati e oppressi quando non beneficiari direttamente di quella o di altra promozione o occasione di crescita professionale. Noi dovremmo, al contrario, favorire la crescita di un sentimento comunitario: vi faceva riferimento molto bene prima la senatrice Fucksia; noi dovremmo lavorare perché proprio il luogo e l'ambiente di lavoro come comunità come comunità diventino il contesto più idoneo nel quale, da un lato, siano di per sé difficili le anomalie, le patologie e i reati che possono essere commessi e, dall'altro, sia più presente un controllo sociale in tutti coloro che concorrono a quell'attività. Nelle pubbliche amministrazioni già oggi vi sono tutele e presidi dedicati alla segnalazione di irregolarità. Soprattutto, occorrerebbe una maggiore iniziativa dello stesso Ministro della pubblica amministrazione, perché ulteriori linee guida possono concorrere a creare quel contesto più escludente le attività patologiche. Il dialogo sociale si è svolto soltanto si è svolto soltanto in relazione al contratto nazionale e per anni, come sappiamo, è rimasto Noi avremmo invece bisogno di un dialogo sociale più diffuso nelle stesse pubbliche amministrazioni, attraverso il quale arrivare a una maturazione delle forme sindacali, che troppo spesso assumono caratteristiche corporative proprio per l'assenza del buon datore di lavoro. Io non parto mai dalla critica al sindacato: esso è normalmente lo specchio del suo datore di lavoro; è il riflesso della qualità del suo datore di lavoro. molto spesso anche i comportamenti sindacali hanno un carattere corporativo, talora perfino non trasparente, ma il dovere delle amministrazioni dovrebbe essere invece quello di favorire un dialogo sociale articolato ambiente per ambiente di lavoro, perché le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad una rivoluzione. Se noi consideriamo banche e assicurazioni, che da sempre sono considerate le attività economiche private più prossime ai modelli organizzativi delle pubbliche amministrazioni, vediamo come le tecnologie digitali abbiano rivoluzionato il modo di lavoro in quegli ambienti, ma non abbiano sostanzialmente cambiato il modo di lavorare nelle pubbliche amministrazioni. Recentemente si discute di un maxiconcorso semplicemente assumendo la linea del *turnover*, cioè del ricambio di coloro che ne escono, mentre invece occorrerebbe una fortissima reingegnerizzazione dei processi e, prima ancora, delle funzioni. Cosa che non è accaduta con la terza rivoluzione industriale, quella dell'informatica. Quindi la digitalizzazione è un'occasione straordinaria ai fini della trasparenza. Io credo nel potere della tecnologia ai fini di trasparenza degli atti; pensando, attraverso la fatturazione elettronica, anche tra privati e privati, e non soltanto nel rapporto tra essi e le pubbliche amministrazioni. Pensiamo che, più in generale, dovremo sempre più smaterializzare gli atti e quindi poter tracciare i comportamenti nel pubblico come nel privato. Quindi anche la tecnologia rappresenta una deterrenza importante rispetto alle anomalie. La legge La legge dovrebbe essere al più in queste materie una *soft law*, una regolazione leggera con rinvio alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e con con rinvio alle responsabilità del Ministro della pubblica amministrazione per i suoi poteri d'indirizzo nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni!

Non dimentichiamo che, se non vi fosse stato l'intervento correttivo della Commissione, si ipotizzava addirittura la buona fede come motivo giustificante la segnalazione infondata: si arrivava a ritenere una indefinibile buona fede come motivo esimente della responsabilità del segnalante temerario

che tutti i danni di quella segnalazione infondata si sono prodotti; danni che nessuno potrebbe poi più recuperare, ma questo ci ricondurrebbe a riflessioni più generali sul nostro sistema giudiziario,

fornisce una protezione generale e astratta e che quindi, per più versi, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Cioè il dipendente segnalante, per potersi sentire veramente tutelato, deve poter far affidamento su una protezione effettiva ed efficace effettiva ed efficace ai fini di contrastare fenomeni di corruzione e di mala amministrazione. Pertanto, la modifica dell'articolo 54-*bis*,

con il decreto-legge n. 90 del 2014 l'ANAC era stata investita di compiti e di responsabilità precise, che erano proprio quelle di disciplinare le procedure. ANAC adempie con queste linee guida che vogliono

Io stessa presentai un disegno di legge nel quale, affidandomi a quella che ritengo sia la migliore pratica per la costruzione delle leggi, leggi, ho cercato di raccogliere e di dare sistematicità alle indicazioni presenti nelle linee guida dell'ANAC, così come credo che dovrebbe fare un buon legislatore: partire dalle buone pratiche e dalle osservazioni che derivano dalla concreta osservazione osservazione di ciò che una legge troppo generica ha posto come premessa, e poi dare una formulazione che renda quella stessa legge più efficiente e quindi più tutelante e corrispondente ai suoi principi.

all'atto della presentazione dei miei emendamenti, credo sia importante richiamare due principi per rispondere anche ad una serie di questioni che sono state sollevate.

è evidente che l'opera di prevenzione è distinta dall'opera di repressione. Così come è evidente che colui che ha in mano tutti gli strumenti per poter fare una denuncia

- nessuno sta toccando. Tutto ciò che è previsto per coloro che intendano denunciare - si tratti anche del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che hanno, peraltro, questo dovere - e tutto ciò che è nella facoltà di qualunque cittadino,

sono uno specifico patrimonio, un modo di pensare di coloro che sono puliti. Noi dobbiamo immaginare che la segnalazione sia il il primo strumento di cui beneficia la stessa amministrazione che, in questo modo, può individuare dei passaggi, dei momenti, degli atteggiamenti, degli inizi di una mala amministrazione e, quindi, può, prima prima di tutto, correggerli. Questa è l'opera di prevenzione. Questa è l'opera fondamentale di prevenzione per la quale tutti noi come legislatori, l'autorità giudiziaria e anche l'Esecutivo chiamiamo in causa l'aiuto, la collaborazione e il senso di responsabilità di ogni singolo cittadino che, con questo provvedimento, viene tutelato proprio nell'esercizio pulito del suo senso del suo essere un *civil servant*, del suo mettere al primo posto la buona gestione dell'amministrazione di cui fa parte. parte. Quest'opera di prevenzione deve essere condotta con degli strumenti adeguati. E la prima tutela, come ho già avuto occasione di dire nell'intervento di ieri pomeriggio, verte proprio sul lavoro, proprio sul rispetto della garanzia di non perdere

comportamento di mala amministrazione e segnalarli al responsabile per la prevenzione della corruzione. Io sono abituata a guardare alle parole e lì noi troviamo il responsabile per la prevenzione. Quindi, tutto quel percorso, che viene invocato, di denuncia e di procure è altra cosa. Qui noi stiamo parlando di una prevenzione di mala amministrazione, dando per scontato che un'amministrazione sana beneficia

questo vale ancora di più, Nel privato, ciò che corrode la capacità delle aziende migliori di stare sul mercato sono proprio i fenomeni corruttivi. Quindi, il privato dovrebbe essere il primo a sostenere la validità e il beneficio di una tutela di chi segnala.

che avalla e conosce i meccanismi di mala amministrazione della sua azienda. Così pure è possibile, ed è assolutamente frequente, che il dipendente del privato, che conosce e sa che stanno verificandosi dei meccanismi di mala amministrazione, non abbia il coraggio di denunciarli. Peggio ancora: se l'azienda

che la cultura del merito deve essere accompagnata da un contesto di lavoro ed economico sano. Credo che nelle parole di chi mi ha preceduto ci sia

ad applicare convenzioni e regole europee: l'ultima, la più recente, è sull'antiriciclaggio, ambito nel quale la normativa europea ci chiede di disciplinare le tutele; quindi dobbiamo farlo, lo stiamo facendo ed è il privato, si parla di banche. un'incoerenza politica: ho sentito tutti stracciarsi le vesti per le vicende collegate alle banche. Benissimo, signori: i più importanti *whistleblowers*,

C'è incoerenza anche rispetto all'economia, per quanto dicevo prima, e credo derivi da un dato antropologico: in questa legislatura, in questo Senato, evidentemente non siamo ancora arrivati a comprendere che la soluzione per l'Italia è la democratizzazione anche della responsabilità della salute del nostro Paese rispetto ai fenomeni corruttivi. Credo vi sia una difficoltà antropologica nel vedere che il sottoposto ha la capacità mettere in discussione l'azione del suo sovrapposto,

la necessità di lottare contro la corruzione e, segnatamente, contro chi per interesse personale prende decisioni contrarie al bene pubblico è una cosa che non solo condivido, ma che pratico, in particolare in quest'Aula. ritengo che la cosa vada fatta nel rispetto delle regole, senza trasformare il nostro Paese e i nostri uffici, pubblici e privati, in uno Stato di Polizia e di delazione, dove

Più che giusto e lo condivido pienamente, ma ritengo odioso l'approfittare di posizioni pubbliche per recare danno alla cosa pubblica che si amministra,

violazione delle regole di concorsi pubblici, di gare di appalto e di altre cose di questo genere perché, proprio dove dovrebbe esserci la regolarità e la competizione leale con regole chiare, chiare, specialmente quando le regole sono dettate dallo Stato, ci deve essere una severità nei confronti di chi commette irregolarità. Detto questo, con questo provvedimento, che ha un bellissimo titolo, si sta facendo un'altra cosa. Si sarebbero potuti fare alcuni interventi e alcuni dettagli di queste norme li ritengo anche positivi, ma la cosa importante è che si dà la possibilità a qualunque lavoratore, addirittura temporaneo o di ditte esterne alla pubblica amministrazione, di guadagnarsi

e che avete un riscontro nel Paese perché gli italiani condividono perfettamente ciò che ho detto e che voi dite e, cioè, che la corruzione semplice: sarebbe troppo facile se ci fossero quelli con l'etichetta dei buoni, che dobbiamo tutelare in ogni caso, e quelli con l'etichetta dei cattivi, che dobbiamo massacrare in ogni caso. Così sarebbe molto facile.

in modo generico qualche condotta illecita da parte della pubblica amministrazione sia il buono e che la persona

bastava il sospetto per essere messi al *paredón*, cioè condannati alla pena capitale, guidata dal suddetto personaggio, riprodotto su tante magliette commerciali. Se questa è la giustizia in cui si crede, allora questo provvedimento va bene.

denuncia - per trovarsi tutelato contro qualunque provvedimento. Avete mai sentito parlare del fatto che non c'è molta meritocrazia nella pubblica amministrazione? Si dice, poi si fanno i convegni su questo tema e magari non la si pratica molto.

cercare di fare la differenza tra il lavoratore che non lavora e il lavoratore che si impegna. Dappertutto, e in particolare negli uffici pubblici, un lavoratore che non fa il proprio lavoro,

potrà godere di anni e anni di tutela rispetto alle sue condizioni di lavoro. Pertanto: «meritocrazia, ciao ciao».

inoltre sottolineare che queste misure sono incredibilmente ampie, perché si riferiscono si riferiscono anche ai collaboratori e ai consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. C'è il rischio che questa norma sia estremamente efficace, non per lottare contro la corruzione, ma per impedire alla pubblica amministrazione di lavorare. Cosa succederà

che rendono la pubblica amministrazione incapace di agire. Non si è mai visto un dirigente punito per aver dato in ritardo un'autorizzazione

finestra") *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, credo che i senatori Buemi, Sacconi, Mazzoni e Compagna, intervenuti ieri e oggi, possano farmi credito di una posizione sempre attenta alle ragioni del garantismo liberale, lontana da ogni pulsione giustizialista. Mi faccio forte di questo credito per chiedere loro di considerare con attenzione maggiore di quanto appare dai loro interventi il contenuto effettivo del disegno di legge Mi sembra, del resto, che i dibattiti di ieri e di questa mattina abbiano fatto registrare molta superficialità da entrambe le parti: sia da parte di chi ha voluto presentare questo disegno di legge come una sorta di incitamento istituzionale alla delazione diffamatoria o come un attentato alla libertà di impresa; sia da parte di chi lo ha presentato come una sorta di panacea, capace di ripulire magicamente il nostro Paese da ogni forma di corruzione. Questo disegno di legge non è né una cosa, né l'altra. Al senatore Malan, che ieri ha parlato di attentato alla libertà di impresa, faccio osservare che, al contrario, l'articolo 2 del disegno di legge è posto proprio a protezione dell'impresa costituita in forma societaria, contro il rischio delle pesanti sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001 conseguenti a episodi di corruzione di cui siano responsabili suoi dirigenti o impiegati. Dice infatti la norma: se doterai la tua struttura aziendale della strumentazione che qui indichiamo per prevenire e contrastare le malversazioni, cioè di almeno un organo-filtro capace di raccogliere e vagliare le segnalazioni di irregolarità provenienti attraverso il canale protetto che qui è indicato, tu società non sarai tenuta responsabile sul piano amministrativo per i reati eventualmente commessi dai tuoi dipendenti. Quale attentato alla libertà di impresa? Al contrario, è una misura posta a tutela dell'impresa sana e corretta. In che cosa consiste l'organo-filtro che il disegno di legge prevede? Si tratta di uno strumento che noi riprendiamo dagli ordinamenti di Paesi che sono altrettante culle dello Stato di diritto e delle libertà individuali: il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America. Altro che attentato alla libertà e ritorno allo Stato di polizia di cui hanno parlato ieri i senatori Sacconi, Compagna e Mazzoni! Questo è uno strumento che è stato utilmente attivato anche per Expo 2015 a Milano, senza dar luogo ad alcuna deriva poliziesca né ad alcun eccesso delatorio, e invece contribuendo efficacemente a prevenire le malversazioni. Per capire di che cosa si tratta, invito i colleghi a mettersi nei panni del dipendente di un'impresa o di un'amministrazione che, per ragione dello svolgimento del suo lavoro, è venuto a conoscenza di qualcosa che gli sembra pericolosamente irregolare: ad esempio la violazione di una procedura aziendale da parte di un ufficio acquisti (faccio solo un esempio). Può essere che si sia trattato soltanto di un'irregolarità isolata, senza dolo e senza danno, ma può essere anche che dietro di essa si nasconda una malversazione grave. Che cosa può fare il nostro dipendente o anche collaboratore? Presentare una denuncia all'autorità giudiziaria? Se poi risulta che non c'è un reato, ciò potrebbe configurare una mancanza anche grave nei confronti dell'impresa datrice di lavoro o dell'amministrazione, persino un reato di violazione di segreto professionale o aziendale. Parlarne con un dirigente dell'impresa? Ma quale dirigente? E se poi quello fosse colluso o compiacente con il malversatore? E, poi, come fare per non mettersi in cattiva luce come ficcanaso importuno? La buona pratica che la nuova norma indica alle imprese - ripeto: sulla scorta delle migliori esperienze internazionali su questo terreno consiste innanzitutto nel dotare la propria struttura di un organo deputato a ricevere qualsiasi segnalazione di questo genere, vagliarne la fondatezza e le implicazioni, archiviarla se la si ritiene non significativa, dare corso alle necessarie indagini se invece si ravvisa un pericolo di malversazione. La buona pratica consiste inoltre nell'attivare almeno un canale di comunicazione riservata per il dipendente, collaboratore o anche soggetto terzo, che gli consenta di compiere la segnalazione con la certezza che essa sarà ricevuta da chi è in grado di valutarne il peso e da chi garantisce di farne solo un buon uso. Nessun "regolamento di conti", dunque, collega Buemi. Nessun anonimato, collega Fucksia. Al contrario, questa buona pratica serve proprio per eliminare ogni possibile ragione per la lettera anonima, proteggendo il nome di chi, assumendosi le proprie responsabilità, collabora a prevenire o scoprire la malversazione e, per altro verso, tutelandolo contro discriminazioni o rappresaglie. Mi rivolgo, a questo proposito, al collega Malan, e lo avevo già sottolineato sottolineato nel mio intervento di ieri: questa tutela non è altro che una specificazione di un divieto di discriminazione e rappresaglia che costituisce già principio generale del nostro ordinamento. Per questo aspetto la legge non aggiunge niente a quanto già potrebbe essere applicato in virtù dell'articolo 15 dello Statuto dei lavoratori. In assenza di questo organo-filtro e di questo canale di comunicazione riservato, che cosa potrebbe e dovrebbe fare la persona in questione? Sarà corretto comunicare la notizia a un dirigente con cui c'è maggiore dimestichezza o invece a terzi? E a quali terzi? In quest'ultimo caso, non c'è il rischio di incorrere nel reato di diffamazione o calunnia, o di violazione del segreto professionale o d'ufficio? E ancora: qual è il limite E se poi le ipotesi tratte dalle informazioni comunicate risultano infondate, o le informazioni stesse irrilevanti? Ci sarà il rischio di conseguenze negative per chi comunica le Oggi il nostro ordinamento non indica con chiarezza che cosa debba fare chi si trovi in questa difficile e scomoda situazione, con la conseguenza che ne risulta incentivato il silenzio dettato da una malintesa prudenza, anche quando l'intenzione della persona in questione non sarebbe l'omertà. L'articolo 622 del codice penale stabilisce che: «Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa (...) è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione ecc.». È molto importante mettere a fuoco lo snodo cruciale di questa disposizione: quello della giusta causa di rivelazione, che si applica non soltanto al segreto professionale,

pubblici). Si tratta, in sostanza, di un principio di bilanciamento tra gli interessi contrapposti, dove però l'ordinamento attuale lascia una zona di indeterminatezza, una zona grigia. Il bilanciamento tra questi interessi in alcuni casi è davvero difficile; e da questo bilanciamento dipende una responsabilità penale del dipendente pubblico o privato che riveli vicende riservate dell'impresa o dell'amministrazione. Il

aggiuntivo. In tutto questo, di poliziesco non vedo proprio nulla. Mentre ci vedo un passo avanti nella direzione dell'allineamento del nostro Paese con quelli all'avanguardia nel coltivare le *civic attitudes*, il senso civico diffuso e radicato. Ne abbiamo bisogno!

«Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23».

infatti, che qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni, ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria. A tal proposito, sorgono delle domande. Dove sono le procedure?

la difficile questione del reintegro, che chiaramente implica il ricorso al giudice del lavoro. Ma chi, di fatto, mette nelle mani del giudice del lavoro la qualifica

Credo che tutti possano immaginare che il datore di lavoro che licenzia non scriverà mai che il licenziamento è dovuto a una segnalazione.

l'operazione - secondo me doverosa - di equiparare tutte le misure che riguardano il dipendente di una pubblica amministrazione e di tutte le altre categorie identificate come tali a quelle

ci si riferisca al fatto specifico. Uno degli aspetti gravemente negativi del testo al nostro esame è che esso più che le segnalazioni, ovvero le denunce circostanziate, incoraggia proprio quelle non circostanziate. Una denuncia,

allora che già oggi nella pubblica amministrazione c'è il problema della quasi impossibilità di promuovere il merito.

i buoni avevano il cappello bianco e i cattivi il cappello nero. Nella realtà però non funziona così. Nella realtà succede che un lavoratore che dovrebbe fare il suo lavoro non lo fa; succede che chi fa una denuncia sia in buona fede e succede che il denunciato

si devono punire i reati quando avvengono; bisogna punire chi commette il reato, anche se occorre tutelare chi fornisce prove per il reato. Non si può però mettere in mano a chiunque un'arma pesantissima che, contemporaneamente, tutela se stessi e danneggia gravemente la pubblica amministrazione.

e, dunque che non ci sia una segnalazione generica. Ripeto che il Gruppo di Forza Italia ed io siamo perfettamente d'accordo nel tutelare chi segnala reati o condotte illecite nella pubblica amministrazione.

a una società, che diversamente non avrebbe incassato, e da quattro anni sono in attesa di sapere chi, presso il Ministero dei trasporti, abbia messo quella firma. Ho provato con l'interrogazione parlamentare; ho provato con l'accesso agli atti di cui alla legge n. 241 del 1990; ho provato con la legge Madia, sempre un muro di gomma. Cosa mi date in cambio ai sensi di questa legge? Bisogna incentivare chi porta prove e non chi fa semplice maldicenza, che non c'è bisogno di incentivare. Basterebbe aver

Ma se invece uno ha fatto accuse generiche, senza fornire elementi di prova, tutela se stesso, danneggia l'amministrazione di cui fa parte, e la collettività, esattamente come se avesse tenuto se avesse tenuto un comportamento contrario alla pubblica amministrazione, che è ciò che si vuole punire. Almeno chiediamo di fornire elementi di prova. Non lasciamo una norma così generica che - ripeto - incita anche chi abbia elementi di prova

approfondimento anche degli esposti, tant'è vero che ancora non c'è nulla di concreto, pur essendoci danni per miliardi alla cosa pubblica. io ho fornito degli elementi concreti. Invece conviene fornire elementi vaghi che, se respingete questo emendamento, confermate, perché non ci saranno alcune possibilità di sanzione e un intervento per stabilire dov'è la realtà e nel frattempo la collettività

il capo di gabinetto del tempo con più funzioni, sia di controllore che di controllato, sulla quale francamente è stato steso

ho risposto sia ieri sia oggi, mi sembra in modo piuttosto compiuto, alla sua critica, osservando sulla tutela antidiscriminatoria come non sia affatto vero che il presente disegno di legge istituisca una protezione automatica e indiscriminata per chiunque faccia una segnalazione. Il disegno di legge in discussione non fa altro che specificare che chi compie una segnalazione è protetto dalla stessa tutela antidiscriminatoria che si applica in generale; la quale non è affatto indiscriminata, perché è rivolta soltanto contro atti di rappresaglia, cioè mirati a punire il fatto di aver segnalato; il che significa che invece tutti i provvedimenti di trasferimento e anche di licenziamento non motivati da rappresaglia vengono trattati esattamente esattamente come nei confronti di tutti gli altri dipendenti dell'azienda o dell'ente pubblico. Quanto al venticello della

che la segnalazione deve essere fatta a un organo-filtro, cioè alla persona specificamente deputata a verificare la fondatezza e la rilevanza di quanto segnalato. Ciò significa che può può avere un senso anche segnalare qualcosa che presenta l'apparenza dell'irregolarità, anche se non c'è una compiuta evidenza della irregolarità stessa e del danno che può derivarne. Tuttavia, proprio il fatto che questa segnalazione avviene in via

non voglio che da questa segnalazione derivi alcun danno alla società o alla singola persona, ma chiedo che chi è competente verifichi. Questo è il contrario della delazione maliziosa o della calunnia; e la funzione dell'organo-filtro è proprio quella che garantisce un trattamento adeguato della segnalazione stessa. Può essere che quello che dico non sia vero, che il disegno di legge non dica questo, non abbia questo effetto, ma chiederei al senatore Malan di non ripetere meccanicamente le stesse cose dette ieri senza almeno replicare alle singole argomentazioni e confutazioni che gli sono state state proposte; altrimenti il dibattito in questa sede è perfettamente inutile.

di concreti ed oggettivi elementi, ma non capisco la sua contrarietà. dobbiamo ascoltarci per quanto possibile senza immobilizzarci al ricatto delle parole, perché le parole sono fragili. Se si vuole mantenere lo Stato di diritto, bisogna stare attenti, perché quando si parla politicamente è chiaro che l'avversario dello Stato di diritto

ma non riesco a capire perché, nella difesa dello spirito e dell'impronta di questo disegno di legge, abbia tanta renitenza a far suo quell'elemento di garanzia che aggiungerebbero

che anche il pubblico ministero, per avviare un'azione di accertamento di responsabilità penale, deve essere in possesso di elementi concreti di prove quantomeno presuntive che possano lasciare immaginare o configurare l'ipotesi di una condotta illecita. Consentendo invece ad un qualsiasi pubblico dipendente di far avviare un'azione in sede di autorità anticorruzione o comunque di procura

da una prova quantomeno concreta che questi abbia commesso un fatto illecito. Non comprendo quindi per quale ragione non vi sia anche l'adesione del senatore Ichino su questo argomento, perché mi pare che si vada tutti nella medesima direzione, come diceva il senatore Compagna, ma con due diversi metodi per l'avvio di determinate attività nella pubblica amministrazione.

chiedono al senatore Ichino come mai sia contrario a specificare che si adducano concreti elementi di prova.

il chiacchiericcio e le cose concrete. Vi è poi un'altra differenza: la calunnia della quale si parla nel Barbiere di Siviglia è calunnia in senso generico, non nel senso del reato penale.

quello che, altrimenti, sarebbe normale chiacchiericcio. Il quale, per carità, è fastidioso, ma forse è un po' più fastidiosa una norma che rischia di far andare in carcere qualcuno senza colpa. Introduciamo questo elemento, per favore, anche perché

Ma allora come fa questo segnalante ad essere colpito da un provvedimento? Il comma 1 presuppone che, nonostante vi sia la garanzia dell'anonimato al comma 3, questa garanzia venga violata. E da chi può violata? Dal responsabile dell'anticorruzione, dall'ANAC stessa o dall'autorità giudiziaria. Altrimenti come sarebbe prendere un provvedimento contro questa persona a motivo della segnalazione? Dunque, ciò vuol dire che, in realtà, il collegamento con la segnalazione viene fatto per via automatica, se un dirigente prende un provvedimento nei confronti di un dipendente, di cui non può sapere se abbia fatto una segnalazione,

nell'antica Roma si misero per iscritto le leggi per evitare che chi le applicava le cambiasse a seconda dei casi e in questo anche Hammurabi fece un passo avanti. Se invece vogliamo tornare a prima di Hammurabi, ditelo, perché qui c'è scritto questo: c'è scritto che se un dirigente prende un provvedimento nei confronti di un dipendente senza sapere che questo dipendente aveva fatto una segnalazione nei confronti di colui che prende questa misura, colui che prende la misura di sanzione nei confronti del dipendente può essere punito. Sarebbe interessante capire il funzionamento di questa legge. Ripeto: almeno chiediamo di addurre elementi di prova, perché altrimenti veramente può succedere qualunque cosa. E mi sono dimenticato di presentare un emendamento che chiedesse anche che queste prove non siano già conosciute:

e la segnala al responsabile anticorruzione. Non c'è scritto da nessuna parte che, se la notizia non è decisiva o se è la millesima persona a denunziarla, le tutele non ci sono più. Suggerisco allora, a chi vuole usufruire di questa legge, di prendersi una delle mie interrogazioni

«ho sentito dire che a Roma ci sono stati problemi con la questione di Mafia Capitale, mentre ero in ufficio dovevo consultare un quotidiano e l'ho saputo», lo segnalo e sono tutelato. Insomma, questa è una legge manifesto, ma in quanto tale dovrebbe fermarsi per l'appunto a questo: presenti un disegno di legge, fai una conferenza stampa, ti fai bello e poi però chiudi lì, perché qui siamo in un'Aula legislativa, non in una sala di conferenze stampa.

Qui stiamo determinando effetti giuridici a seguito di una generica segnalazione. Quando si aggiungono i fatti concreti di cui parla il senatore Malan nel suo emendamento, allora quella segnalazione assume i connotati di una denuncia, con tutte le conseguenze eventualmente penalmente rilevanti nel caso in cui quei fatti non fossero accertati o non fossero veri. Con la semplice segnalazione, però, s'introduce nel nostro ordinamento un qualcosa che dà avvio ad un procedimento penale

che clima lavorativo creerà nelle nostre imprese, pubbliche e private? Sarà uno *stress* allucinante. Vi è poi un altro fatto. Tutti sanno quali sono la mia stima e il mio affetto nei confronti del senatore Ichino,

che anche queste strutture, nominate magari dal datore di lavoro o da chiunque, possano avere secondi fini o essere utilizzate per fare segnalazioni preferenziali e delle esclusioni.

brevemente per dire che il cittadino, il dipendente, l'impiegato o il collaboratore non è un pubblico ministero. Non gli si può accollare l'onere di un'indagine compiuta su tutto quanto emerge. Per altro verso, nei Paesi civili è considerato utile per la prevenzione della malversazione qualsiasi informazione su irregolarità che possano essere o anche non essere la punta dell'*iceberg* del reato. Lo strumento che stiamo delineando serve proprio a consentire che la notizia arrivi a chi di dovere; e non nella forma scandalistica

calunnia, alla diffamazione o alle rivelazioni di segreto aziendale o d'ufficio; mentre la segnalazione compiuta correttamente nella forma che non può causare danni collaterali, e che offre a chi dovere lo strumento per la verifica, viene privilegiata ed è indicata al cittadino dotato di senso civico come il modo corretto per informare chi di dovere. Questo è il motivo per cui è sbagliato porre a carico del cittadino che segnala l'onere di costruire un'accusa

a un uso improprio e degenerato anche di questo meccanismo, qualora il disegno di legge diventasse legge. Ve lo immaginate un dipendente pubblico infedele, con il sospetto di essere in una condizione di potenziale trasferimento

azione di rimozione o di verifica ulteriore? Basta che faccia la segnalazione e si mette al riparo da qualsiasi cosa. Il suo dirigente può anche essere colluso con altri ambienti, ma magari sul fatto specifico riguardante il dipendente denunciante può avere ragione perché ci sono elementi di necessità positiva per rimuovere quel dipendente. I giornali di oggi parlano di due ville in un parco pubblico o in un luogo in cui non ci dovevano essere, a Roma. Ho sentito alcune interviste in televisione di pubblici funzionari di un municipio di Roma rispetto alla mancanza assoluta di opere di urbanizzazione in quartieri

dentro le quali guazza un po' di tutto. E allora noi cosa facciamo? Diamo la possibilità di mettersi al riparo semplicemente con una segnalazione generica, che poi spetta ad altri accertare. Credo che, invece, occorra un'assunzione di responsabilità precisa, come ho detto nel mio intervento in discussione generale: c'è in questo Paese gente onesta, che si assume la responsabilità della segnalazione, perché questo è un dovere civico e non deve essere protetto da provvedimenti di particolare privilegio, che inducono comportamenti perversi. di diritto ha bisogno di norme chiare, che responsabilizzino. Abbiamo una stampa che riteniamo libera, che ha possibilità di fare inchieste, se c'è qualcuno che deve segnalare qualcosa e ha paura di ritorsioni ne parli con la stampa; la stampa fa tante inchieste banali, inchieste banali, va a intervistare sul colore delle mutande di qualcuno e invece non si occupa di cose che riguardano la pubblica amministrazione, per le quali ci sarebbero argomenti da vendere in tutta Italia. Poi, colleghi, ribadisco: è ora che introduciamo nuovamente i controlli preventivi sugli atti della pubblica amministrazione,

Vorrei segnalare questo emendamento come indicativo di come dovrebbe essere l'Italia a «cinque

al di là delle intenzioni del legislatore, non determini qualche problema all'interno della pubblica amministrazione.

Però, rispetto al testo della Camera, sono stati eliminati sia

se io, per fregarla, mi rivolgessi a un qualsiasi dipendente della pubblica amministrazione (non a un dipendente del Senato) e gli facessi arrivare una notizia secondo cui il senatore Ichino sta trattando, in ragione di una norma, determinati vantaggi.

quello ha fatto la segnalazione, siccome la notizia è generica e non deve essere una notizia vestita, che cosa avviene? Noi blocchiamo gran parte dell'attività dall'ANAC e degli organi disciplinari. Sarebbe

proprio ufficio; basta vedere le statistiche dei reati contro la pubblica amministrazione, che dimostrano che questa enorme situazione di illecito non c'è.

Non costerà nulla scrivere all'ANAC o agli organi disciplinari, i quali dovranno svolgere un'attività amministrativa anche se la notizia è completamente infondata, sia pure solo per archiviarla.

debba svolgere un accertamento ma quanto meno valutare se è proprio destituita di qualsiasi fondamento, se si tratta di un'attività di *gossip* o addirittura se si tratta di un'attività di terzi che fanno veicolare notizie false.

Ci rendiamo conto che stiamo approvando una norma che nella sua attuazione sarà un disastro e che addirittura determinerà l'inefficienza degli organi che abbiamo creato per combattere la corruzione?

almeno sotto il profilo dell'efficienza complessiva del sistema, la segnalazione. Se invece lasciamo la norma così com'è, senatore Ichino, non troviamo più giustificazione. Capisco tutto quello che lei ha detto prima, ma è difficile

il risultato finale, quale sarà l'effetto di una determinata previsione. Per questa ragione, credo che il voto favorevole a questo emendamento garantisca una vera attuazione delle finalità della norma. Se invece si vuole fare soltanto propaganda, fate pure, perché tra l'altro questa norma, scritta così, non avrà effetto, ma determinerà situazioni di inattività nell'ANAC e negli organi disciplinari. in buona sostanza, riassumendo l'intervento del senatore Caliendo, noi chiediamo semplicemente che si realizzi in maniera chiara un coordinamento tra le norme penali in tema di tutela della onorabilità

Perché mai per altri vi è l'ipotesi del delitto di calunnia e di diffamazione e per il sussurratore - perché qui si tratta di sussurrare

pesantemente sanzionati, debbano per lo meno essere successivi alla segnalazione da parte del dipendente. Mi spiego meglio: si parte sempre dal giusto proposito di proteggere chi segnala fatti contrari all'interesse pubblico e fatti illeciti e si vuole evitare che chi segnala tali fatti venga sottoposto a sanzioni.

rischia una sanzione minima di 5.000 euro. Ma stiamo scherzando? Il dirigente di un ufficio, che è assolutamente certo della sua buona fede e della sua buona condotta, sa che ha sempre fatto tutto - e devo dire che, con tutti gli adempimenti burocratici

non può a cuor leggero prendere provvedimenti organizzativi che possono vagamente danneggiare qualcuno perché se uno di coloro che sono colpiti dal suo provvedimento ha fatto una segnalazione contro altri, magari una persona che lo stesso dirigente disprezza e che teme tenga comportamenti scorretti, il dirigente viene colpito con la sanzione da 5.000 euro in su.

modo si paralizza la pubblica amministrazione. Già oggi è molto difficile prendere provvedimenti di qualunque tipo che riguardano l'organizzazione dei lavoratori, e in parte è un'ottima cosa perché bisogna tutelare i lavoratori in generale, che facciano o meno segnalazioni. siccome siamo nel mondo della realtà e ci sono lavoratori che si comportano male accanto ad altri che si comportano bene - i quali, dunque, subiscono due volte le conseguenze del comportamento di quelli che si comportano male, in altre parole che non lavorano

rischia una sanzione da 5.000 euro in su. Questo è ciò di cui stiamo parlando. Ecco perché chiedo che, almeno secondo una vaga logica, la decisione debba essere successiva,

che c'è un provvedimento che potrebbe danneggiarlo - il dirigente viene colpito dalla sanzione di 5.000 euro. Ma veramente? Era difficile scrivere una norma peggiore di

che riguarda una disciplina particolare delle aziende private. La struttura del provvedimento è veramente di rara irrazionalità. Volevo usare una parola più pesante, ma mi sembra corretto usare questa. *(Applausi dal

Ma vi rendete conto che state mortificando il diritto di difesa? Per potersi difendere, l'incolpato ha necessità di conoscere le generalità del sussurratore, non lo può conoscere, o - meglio - può sapere chi è soltanto se chi lo incolpa presta consenso a dichiarare la sua identità. Voi non vi rendete conto

provvedimenti, perché rischiamo di compromettere la nostra storia del diritto e la civiltà giuridica che ci viene riconosciuta a livello mondiale.

In conseguenza di queste caratteristiche dell'ufficio pubblico si manifestano intensamente, purtroppo, atteggiamenti che muovono da sentimenti non nobili, come l'invidia e la gelosia. Se c'è un'evidente necessità nelle funzioni pubbliche, è quella di irrobustire la gerarchia e non di indebolirla. Abbiamo bisogno di spirito di comunità, per un verso, ma anche di gerarchia, per un altro.

ma che non siamo mai riusciti a rendere effettiva, anche perché fortemente condizionata dai molti meccanismi delegittimanti o inibenti l'assunzione di responsabilità dirigenziali. Attraverso questo provvedimento ad inibire tale responsabilità, impaurire il dirigente, non mettendolo nelle condizioni di fare ciò che è giusto per il funzionamento di quell'ufficio, compresi i provvedimenti sanzionatori che nelle amministrazioni pubbliche sono rari e, ove adottati, si risolvono quasi sempre in danno di chi li adotta e non di chi dovrebbe esserne spesso il giustificato destinatario.

populiste del Movimento 5 Stelle, perché a non seguirle sembra che uno sta dall'altra parte, con i corrotti. Ciò non è assolutamente vero. C'è un limite a tutto, un limite di ragionevolezza che sarebbe bene che uno Stato di diritto non oltrepassasse mai.

e, cioè, che perlomeno le misure organizzative di carattere generale di un'azienda pubblica, di un ufficio pubblico,

reato. Sarebbe assurdo che non si possa riorganizzare un ufficio, una struttura pubblica, se uno dei dipendenti di questa struttura avesse fatto una segnalazione. C'è sempre il problema che segnalo, e su cui non ho risposte: se il comma 3 garantisce la inconoscibilità dell'identità del segnalante, come fa il dirigente, o comunque il responsabile, a prevenire le proprie azioni a svantaggio di quella persona? I casi sono due:

(e mi risulta che norme giuridiche di carattere generale ce lo dovrebbero dire). Dunque, ciò significa che questa norma è perfettamente inutile e totalmente inapplicabile. Infatti, se non si può conoscere l'identità del segnalante ed è reato solo quando si prendono provvedimenti, che poi vengono definiti ritorsivi, solo quando tu sai che la persona è un segnalante, allora vuol dire che la norma non si applica mai. Questa è logica; bisognerebbe anche applicare la logica, oltre a cercare di apparire sui *media* come grandi combattenti contro la corruzione. Forse anche perché nei Comuni

Pertanto, direi che non ci siamo. Se però la norma si applica anche nel caso in cui non si sappia che una delle persone

allora la conseguenza è che mai un dirigente prenderà un provvedimento qualsiasi che crei qualsivoglia tipo di disagio, come dice il comma 1 (non è che lo sto inventando a tutti coloro che lavorano sotto la propria responsabilità, per timore di essere soggetto a una sanzione da 5.000 euro in su. Dirò di più. In particolare, il dirigente si asterrà dal farlo nei confronti di una persona particolarmente riottosa a fare il proprio dovere.

Stato, queste persone sarebbero proprio quelle che immediatamente si tutelerebbero facendo una qualche segnalazione generica. Sarebbe una cosa matematica. È ovvio che non tutti coloro che segnalano illeciti nella pubblica amministrazione siano cattivi lavoratori; anzi, probabilmente coloro che lo fanno in buona fede e fornendo prove sono anche migliori come lavoratori, e proprio perché sono bravi lavoratori, sono particolarmente indignati per i fenomeni illeciti che avvengono nella pubblica amministrazione.

Quello che però è sicuro è che un cattivo lavoratore con un po' di sale in zucca provvederà a fare una segnalazione, perché così sarà tutelato. Questa è una certezza. Dunque, il dirigente che debba prendere provvedimenti, non prenderà alcun provvedimento che crei qualunque tipo di disagio a uno dei suoi dipendenti, ma soprattutto non lo farà mai nei confronti di un lavoratore riottoso a compiere il suo dovere, e cioè che lo direbbero i moralisti - ruba lo stipendio, vive sulle spalle degli italiani. Però gli diamo la tutela e il salvacondotto con una legge che forse è scritta abbastanza male da essere inapplicabile, ma io non mi fiderei troppo. Tanto meno mi fiderei

non compie il proprio dovere subisca almeno qualche conseguenza negativa. Questa persona non lo farà, perché temerà di prendere multe da 5.000 euro in su, cosa che evidentemente una persona normale non fa certamente a cuor leggero, può venire una multa da 5.000 euro, ma possono esserci tanti episodi e magari c'è più di una persona che ha fatto queste segnalazioni; di conseguenza, fare il dirigente pubblico che cerca di fare il proprio dovere diventerà una cosa da ricchi, ma molto ricchi, e non si vede perché

perlomeno degli emendamenti, ma visto come stanno andando le cose temo che ciò non potrà accadere nella mattinata di oggi. Propongo pertanto all'Assemblea di concludere anticipatamente i nostri lavori alle ore 12,30

Presidente, ci opponiamo a questa richiesta perché è evidente l'intento ostruzionistico da parte del Gruppo Forza Italia-Il

ciò avverrà o se invece dovranno sottostare a un ricatto sulla legge elettorale, perché questa possa passare al Senato con i voti di Forza Italia e della Lega Presidente, vorrei dire che ero in dubbio sulla richiesta del senatore Calderoli, ma ho ascoltato adesso il senatore Crimi parlare di ricatto e io non accetto che le questioni vengano poste su questo piano, quindi accolgo la richiesta del senatore Calderoli.

Signora Presidente, secondo lei è giusto che una persona scelga di morire perché non riceve l'assistenza sanitaria? Parlo di un invalido grave, paraplegico e cieco, ma che vorrebbe vivere, che avrebbe diritto a vivere. Le parlo del Veneto, che è una Regione in cui chi amministra la sanità dichiara che è una delle migliori del mondo, ma forse lo dichiarano solo loro. Questa è la storia di Loris Bertocco, pubblicata oggi in prima pagina su «la Repubblica» e probabilmente la conosciamo tutti. Mi chiedo e le chiedo, signora Presidente, se ha la cortesia di ascoltarmi, se può considerarsi se può considerarsi civile un Paese che nega l'assistenza sanitaria a chi più di chiunque altro ne avrebbe bisogno,

Considerata la drammaticità e l'urgenza di questa situazione, che riguarda la mancata o insufficiente assistenza a tutti i disabili gravi che non dispongono di risorse proprie per assicurarsi le cure necessarie e per condurre una vita dignitosa, chiedo al Presidente chiedo al Presidente del Senato, di farsi parte attiva per rappresentare al Presidente della Regione Veneto la preoccupazione di questa Istituzione rispetto alla più grave delle violazioni di diritti umani,

Signora Presidente, vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea l'ennesimo tentativo di difendere l'interesse di pochi a scapito della salute di molti. Non è certamente l'unico caso in Italia, ma lo riporto perché sta avvenendo in questo momento.

perché il metodo non va bene. E non solo: un dirigente della ULSS si permette di tirare di tirare già le conclusioni. L'organo che dovrebbe tutelare la nostra salute e, per farlo, dovrebbe compiere queste indagini (e infatti ne propone un'altra) anticipa le conclusioni, dicendo che non c'è alcun problema. La fabbrica inquinante che si pensa causi problemi non ha alcuna rilevanza e la ULSS, testualmente, dice che «dà un contributo modesto, se non nullo». Come può permettersi il dottor Cinquetti della ULSS di Treviso di tirare già le conclusioni se non sono stati condotti gli studi? condotti gli studi? E il sindaco, purtroppo, si piega alla volontà della ULSS. Ora, la fabbrica in questione non è una fabbrica normale ma un cementificio, che da vent'anni brucia i copertoni anni brucia il *pet coke*, il peggio del peggio del petrolio. E adesso si vorrebbe farle bruciare anche la plastica: materiali assolutamente innocui da bruciare. Questo è l'ennesimo caso in cui la politica, che ha voce in capitolo

molto veloce, in sei mesi, ed economico. Invece, ne farà fare uno alla ULSS che durerà dieci anni; pertanto, le risposte le avremo tra dieci anni. Questa non è la maniera di tutelare la salute di una popolazione.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, ai nostri figli occorre insegnare la gioia e la speranza. Bambini e bambine, ragazze e ragazzi, hanno diritto alla spensieratezza, al divertimento, al gioco e perfino all'errore. Però, signora Presidente, questi non sono i tempi migliori per coltivare la leggerezza d'animo e l'allegria.

nell'organizzazione di una pretesa marcia su Roma il 28 ottobre. Una rievocazione tragica degli eventi che condussero al ventennio, alla eliminazione degli oppositori, alle leggi razziali e alla guerra mondiale. Per fortuna, la Questura di Roma ha già fatto sapere che non risulta pervenuto alcun preavviso di ordine pubblico e che se pervenisse la manifestazione verrebbe vietata. Signora Presidente, le leggi devono essere però applicate e ve ne sono diverse che vietano l'apologia di reato, l'istigazione a delinquere, la ricostituzione del Partito fascista. Queste leggi non sono applicate con il dovuto rigore.